L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Al di là degli annunci del nostro Presidente del Consiglio, che si sforza di sviare le attenzioni andando in Europa a dire che, per chiudere gli accordi con la Turchia, bisogna mettere a disposizione anche parte di quello che sta riguardando il sistema di informazione della Turchia, vorrei denunciare le purghe da tipico regime attuate oggi all'interno della RAI. Vorrei che ci fosse una maggiore attenzione vorrei capire come la Commissione di vigilanza intenda intervenire, perché ormai siamo alle invasioni barbariche all'interno del nostro sistema di informazione. nel silenzio che anima quest'Assemblea (quando in altri momenti gli intellettuali della sinistra si mobilitavano), se oggi questa attenzione deve cadere e se dobbiamo far continuare lo scempio che si sta perpetrando nella RAI. *(Applausi

di giudice tavolare della zona del Friuli-Venezia Giulia, per i quali avevamo indicato quello che correttamente il senatore Zeller ripropone e che quindi voto con piacere.

di volontaria giurisdizione e un altro. Un giorno lontano forse il senatore Cucca lo spiegherà ai dottrinari che valuteranno la bontà di questo provvedimento.

se i colleghi avessero letto bene i due emendamenti, avrebbero notato che, al di là del

i provvedimenti che possono essere delegati al giudice di pace solo a quelli di minore complessità. Poiché siamo in un campo molto delicato, quello del regime immobiliare, assieme

tutti i provvedimenti legati al giudice tavolare al giudice di pace. Per questo motivo i due emendamenti hanno una finalità simile, ma sono assai diversi

dalla norma non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; dall'altro lato, però, l'articolo 8 proposto dalla Commissione si rende ben conto che tutta questa materia non può che creare inevitabilmente variazioni alla finanza pubblica, tanto più che nella legge di stabilità i finanziamenti per la magistratura onoraria sono stati ridotti.

decidere delle variazioni. Credo che questa sia una spiacevole dimostrazione di incoerenza rispetto alla facoltà del Parlamento di agire sul piano legislativo con una certa libertà, anche rispetto alle coperture finanziarie. Signor Presidente, anche noi voteremo contro l'articolo di copertura di questo provvedimento, perché lo riteniamo non in linea con le previsioni che normalmente dovrebbero essere seguite per ottemperare all'articolo 81 della Costituzione. Per quanto vi sia una riserva di indicazione di successive fonti finanziarie, per coprire eventuali maggiori spese, questa riserva non è mai stata introdotta nel nostro ordinamento, perché è sempre stata utilizzata la formula compensativa: molte deleghe sono state fatte nell'ambito delle somme stanziate o ad invarianza di oneri

caso ci troviamo in presenza di una novità, che è la possibilità per il Governo di indicare nei decreti delegati nuove fonti di copertura, il che contrasta palesemente con le nostre norme di bilancio

perché è una prerogativa in più che questo Governo si vuole attribuire, oltre alle tantissime altre che si sta attribuendo al di fuori delle leggi ordinarie e costituzionali, ma anche perché per qualsiasi altro futuro

collide con l'articolo 81 della Costituzione e con tutta la prassi parlamentare. A parte questo, che è comunque sicuramente un *vulnus* da evitarsi (e quindi anche per questo voteremo contro) vi è un altro aspetto

dei decreti saranno sicuramente superiori alle coperture che oggi indica. Questa è una confessione aperta e assolutamente chiara di incapienza delle fonti di copertura della legge. Ma vi è di più: i contenuti di questo provvedimento, così come si stanno evidenziando alla fine del dibattito in Aula, lasciano intravedere in in maniera abbastanza chiara che stiamo creando una categoria di magistrati che, per le condizioni di proroga e di rinnovo dei contratti, per le condizioni di proroga e di rinnovo dei contratti, a breve potranno sicuramente attivare una serie di contenziosi in virtù del diritto del lavoro vigente nel nostro Paese, e soprattutto della giurisprudenza sul diritto del lavoro che ormai è abbastanza consolidata, per ottenere il riconoscimento di dipendenti ordinari dello Stato con tutte le conseguenze di carattere economico che ciò può comportare. Questo per quanto riguarda il carattere economico. In più, nel merito, stiamo attivando una procedura che potrebbe portare ad un incremento dei ranghi della magistratura eludendo le fasi concorsuali. Infatti se ci dovesse essere un riconoscimento attraverso una causa di lavoro dell'inserimento a tempo indeterminato e a tempo pieno di questi magistrati nel corpo della magistratura, ci sarebbe sicuramente un'invasione in quell'ordine giudiziario di magistrati che non hanno espletato alcun concorso.

competenza in Commissione, ma comunque anche di merito per quelle che sono mie personali valutazioni, mi portano a dire che voteremo sicuramente e convintamente contro l'articolo 8. finestra"). Salutiamo docenti e studenti dell'Istituto tecnico statale «Michele Laporta» di Galatina, in provincia di Lecce, che stanno assistendo numerosi ai nostri lavori.

senatore D'Alì in merito all'esecrabile prassi della decretazione delegata finalizzata a trovare le coperture finanziarie, con l'emendamento 8.0.300 - sarà l'ultimo voto che esprimeremo - miriamo a modificare una disposizione dell'ultima legge di stabilità

per il 2017 alla voce indennità sia dei giudici di pace che dei magistrati onorari. Verosimilmente, con queste risorse, qualora tornassero nella disponibilità di quel capitolo di bilancio in caso di approvazione di questo provvedimento, la la necessità di un'eventuale e successiva decretazione delegata ai fini di tutelare l'invarianza finanziaria sarebbe inutile, motivo per il quale annunciamo il voto favorevole del Gruppo, invitando gli altri Gruppi a

dopo diversi anni di proroghe e provvedimenti diciamo frastagliati in tema di magistratura onoraria. L'esigenza di realizzare una figura unica di giudice onorario e, quindi, di sostituire il GOA, il giudice aggregato di tribunale, il giudice di pace con un'unica figura, che in qualche modo venisse regolata da una legge dello Stato, mi è sembrata cosa saggia. Quindi, al di là dei rilievi che pur sono stati mossi nell'ambito dell'esame del provvedimento, la conclusione non può che essere di voto favorevole allo stesso. Certo,

il giudice onorario addetto all'ufficio del giudice, che non ha potere giurisdizionale (nel senso che non può decidere le cause)

giudice, ai sensi del secondo comma dell'articolo 101 della Costituzione, nell'ambito della sua attività giurisdizionale non può che avere l'obbligo di rispettare la legge e non può certamente decidere sulla base di un suggerimento, seppure questo gli venga da un giudice professionale togato. Io mi auguro che questa disposizione, che vede licenziato un provvedimento con un'ombra di incostituzionalità, possa essere migliorata.

è un organo sostanzialmente politico, di politica professionale, con elezioni che vedono contrapposte varie fazioni

della politica, mi pare che ci avviamo verso un sistema, che non è certamente italiano e che non lo è mai stato, di una magistratura assoggettata in qualche modo al potere politico ed esecutivo. Certo, è poca cosa rispetto al pericolo che io prospetto, ma è un piccolo passo che, secondo me, non andrebbe fatto. Sul piano pratico, chi ha immaginato questa disposizione non conosce affatto un giudice di pace che si trova dinanzi a sé una parte rappresentata da un avvocato componente del consiglio dell'ordine, sapendo che quel signor avvocato, dopodomani, dopodomani, dovrà esprimere un parere di favore e di gradevolezza positivo della sua attività professionale. Ora, io faccio muovere tutto, sempre, dall'elemento umano, anche inconsapevolmente. Diceva ieri il Sottosegretario per la giustizia in Aula che noi facciamo le leggi sul presupposto di avere dinanzi persone perbene. Io non ho dubbi che una persona perbene, ancorché il giudice di pace gli dia torto, eventualmente esprimerà su di lui un parere favorevole, anche avendo avuto torto da quel giudice. Ma l'essere perbene non può contrastare con l'elemento umano. Ed è umano che se un giudice, come avvocato, mi dà torto in una causa e poi mi dà torto in un'altra e in un'altra

evitare che una funzione giurisdizionale venisse in qualche modo condizionata da un parere che spesso può nascere sulla base di una emozione umana. Non sono stato ascoltato neanche in questo. Ho cercato di far passare un subemendamento all'emendamento del relatore.

a prescindere dalla soluzione e dalla definizione del procedimento, cioè della richiesta di rinvio a giudizio o della archiviazione. È provocatorio, quel subemendamento. È provocatorio perché il Ministro deve sapere - ed è bene che lo sappia - che, ove mai nel decreto attuativo si dovesse prevedere una diversa indennità per il provvedimento che definisce il giudizio di archiviazione rispetto al provvedimento che definisce il procedimento con la richiesta di rinvio a giudizio, io personalmente farò barricate. Perché non si può immaginare sereno un giudice che sappia che, adottando un provvedimento, incamererà una cifra superiore

Signora Sottosegretaria, non venga in Parlamento con un decreto delegato attuativo che prevede una diversa indennità tra le due diverse ipotesi di definizione del procedimento,

chiedi il proscioglimento incameri dieci, se invece chiedi il rinvio a giudizio incameri cinquanta. E non mi venga a dire che le leggi le facciamo per le persone perbene, perché me la trovi lei una persona perbene che, di come definisce i procedimenti, incamera 5.000 euro al mese o 1.000 euro al mese; trovi lei una persona perbene che rinuncia a 4.000 euro per fare, come dice lei, una sostanziale giustizia. Ciò nonostante, in questa fase, e in attesa di un'attenzione maggiore, sperando che il provvedimento nell'altra Camera abbia un relatore (mi consentirà di dirlo il senatore Cucca, al quale sono molto affezionato)

del Paese ad avere una regolamentazione della magistratura onoraria, che - ahimè - è divenuta il pilastro portante del sistema giustizia italiano. Quindi, per queste ragioni preminenti, esprimeremo un voto favorevole, pur con le critiche che ho appena denunciato.

ci ha pensato il rapporto annuale della Commissione europea per l'efficienza della giustizia a far cadere l'ultimo alibi rispetto alle inefficienze e alla lentezza del nostro sistema giudiziario. Era opinione diffusa, infatti, che dedicassimo poche risorse al sistema giustizia. Così non è. La fotografia della Commissione, che guarda all'anno 2012, dice che il nostro Paese ha investito 4,5 miliardi nel sistema giustizia: terzo, solo dietro a Germania e Regno Unito. Mi preme altresì evidenziare quanto questo costi ad ogni singolo cittadino. alla ricaduta *pro capite* delle risorse destinate da ogni singolo Paese alla giustizia, se la media europea è di 35 euro a persona, in Italia il sistema giudiziario (giudici, pubblici ministeri, personale amministrativo) costa 50 euro a persona, in media. Questo è un onere molto ingente, infatti la Banca d'Italia lo misura nell'1 per cento del PIL: credo che questo sia un dato molto sconfortante rispetto al risultato finale, cioè rispetto al servizio. Le analisi comparative internazionali svolte dalla Banca mondiale hanno confermato che il sistema della giustizia civile costituisce il tallone d'Achille del nostro sistema economico, collocando l'Italia al 158° posto nell'e*nforcing contracts* *rank* (la classifica di esecuzione con una durata media delle procedure di recupero del credito di 1.210 giorni; praticamente tre anni per recuperare un credito. A questo si aggiunga che la media del costo per recuperare il credito è pari al 30 per cento. Insomma, nel settore giustizia siamo riusciti ad elaborare un nuovo modello economico: quello del massimo onere per un minimo risultato. La giustizia - e mi riferisco allo specifico settore di quella civile - ha un'esiziale urgenza di trasformarsi da macigno sull'economia a volano della ripresa economica del nostro Paese. Dopo una lunga stagione di riforme, che molto poco hanno effettivamente riformato, è ormai un imperativo categorico addivenire ad un processo che possa garantire, in ogni fase e grado di giudizio, efficacia e tempestività delle decisioni. È in tale contesto che si colloca il disegno di legge delega oggi in discussione, con il quale il Governo si propone di procedere ad una riforma organica e complessiva della magistratura onoraria, ritenendo non più adeguata l'attuale disciplina della stessa, oggi modulata differentemente a seconda che si tratti di giudici di pace, ovvero di giudici onorari di tribunale e ovviamente di vice procuratori onorari. Tale disegno di legge, che segue numerosi altri di iniziativa parlamentare, persegue il pur condivisibile fine di ridisegnare la magistratura onoraria mediante la predisposizione di uno statuto unico applicabile indifferentemente a tutta la magistratura onoraria. Non solo, il disegno di legge oggi in Aula, interpretando ed attualizzando le previsioni di cui agli articoli 43 e 43*-bis* dell'ordinamento giudiziario, intende anche valorizzare il ruolo dei giudici non togati, emancipandoli dalla mera funzione sostitutiva di giudici impediti o assenti, tramite l'introduzione di tre possibili modelli organizzativi: affiancamento, supplenza ed infine ruolo autonomo. Nel riconoscere, a tale proposito, l'indispensabilità del contributo che la magistratura onoraria quotidianamente offre all'amministrazione della giustizia, soprattutto quella di prossimità, non posso tuttavia esimermi dal fare alcune brevi considerazioni non circoscritte al solo testo in discussione. Esso, con tutte le limitazioni che io e il Gruppo dei Conservatori e Riformisti abbiamo sottolineato con la nostra attività emendativa, pur costituendo un apprezzabile lavoro di rammendo - e sottolineo di rammendo - del logoro tessuto giustizia, purtroppo - è bene dirselo chiaramente - costituisce l'ennesimo tentativo legislativo dal carattere meramente riparatorio, ma di certo non risolutivo di un problema che richiederebbe un radicale mutamento di prospettiva, che transiti per una riorganizzazione sistematica, organica e complessiva del sistema giustizia. altro versante sul quale si potrebbe incidere, nell'ottica dell'efficienza, è quello della riorganizzazione giudiziaria. Sotto questo profilo ritengo che sarebbe auspicabile la soppressione di alcuni uffici: si pensi ai tribunali regionali delle acque pubbliche o alle sezioni specializzate agrarie, le cui attribuzioni sono troppo spesso fonte di questioni e conflitti di competenza delle quali il sistema processuale dovrebbe e potrebbe certamente fare a meno. Sarebbe opportuno, inoltre, un ripensamento delle funzioni magistraturali che transiti dal chiaro riconoscimento, anche sul piano della normazione primaria, delle posizioni professionali dei magistrati ordinari, che si dovrebbero differenziare in ragione della specializzazione funzionale. È chiaro infatti che, a fronte della straordinaria complessità raggiunta dall'attuale quadro normativo, l'esigenza di una specializzazione delle funzioni giudiziarie (magari temperata da criteri temporali di rotazione) e di una efficace suddivisione del lavoro secondo criteri di materie per aree omogenee, rappresenta ormai l'indispensabile presupposto di una giustizia efficiente. Ciò consentirebbe di non disperdere le competenze conseguite e potrebbe contribuire, quale effetto virtuoso dell'elevata conoscenza acquisibile nei singoli campi del sapere giuridico, ad un forte incremento della produttività degli uffici giudiziari ed alla conseguente riduzione dei tempi di definizione delle controversie. non posso esimermi dal segnalare che un altro elemento indispensabile per una seria innovazione della giustizia è quello della riforma dell'avvocatura (ormai non più procrastinabile), che non può più prescindere dall'introduzione di un numero programmato di ingressi nei ranghi della classe forense. L'attuale sistema, infatti, ha contribuito a determinare, con sempre più allarmante frequenza, il fenomeno della cosiddetta domanda anomala di giustizia, ossia di un'abnorme reiterazione di iniziative giudiziarie per questioni di carattere seriale e di modesto valore economico che intasano gli uffici giudiziari di primo grado, impegnando, in modo sproporzionato rispetto all'interesse tutelato, le energie dei giudici e del personale amministrativo e contribuendo in modo determinante alla dilatazione dei tempi medi di durata dei processi. nella medesima direzione è necessaria una radicale modifica del regime del patrocinio a spese dello Stato, spesso concausa del menzionato fenomeno di domanda anomala, otre che di un ingente onere per la collettività. In definitiva, il provvedimento che ci apprestiamo a votare è un tentativo di mettere delle toppe. Purtroppo, i problemi del sistema giustizia non possono essere risolti a *spot*, in quanto sarebbe necessaria una riforma

in linea con quella che è oggi la mentalità del partito di maggioranza relativa: a buoni propositi seguono sempre una serie di soluzioni poco congeniali.

con una proposta che, per certi versi, invita a tirare un sospiro di sollievo quasi per tutti quei magistrati onorari che, comunque, stanno lavorando da anni

i professionisti che hanno sottratto tempo a una propria professione, spesso svolgendo più professioni.

Riusciamo con questa norma ad assicurare l'imparzialità, la terzietà e l'indipendenza del magistrato?

Di sicuro si ha una forma di vantaggio da questo provvedimento perché di certo dà delle garanzie a queste figure di magistrati,

Però, alla fine di tutto non si è certi di poter continuare fino a un'età pensionabile. Dipende dall'età in cui si comincia. Diventa un secondo lavoro. Però, considerare la magistratura un secondo lavoro è quantomeno pericoloso.

Come farà a rispondere per una sua decisione, quando si è attenuto ad una direttiva? Se invece non si fosse attenuto a tale direttiva, per una questione di principio,

non può che essere salutato favorevolmente l'allargamento delle competenze del giudice di pace e della magistratura onoraria, il che porta, evidentemente, ad una riduzione del carico per i giudici ordinari.

di limitazioni di ordine fattuale che costringono a procedere per questa via. Si interviene soprattutto in una serie di materie, che sono poi quelle che prevalentemente intasano i tribunali. Chiunque abbia un po' esperienza in questa materia, finisce per saperlo benissimo: si va dalle questioni condominiali, a quelle successorie, dalla comunione ai diritti reali di varia natura, dai beni mobili (per un valore delle cause che si alza fino a 30.000 euro)

Forse si presta anche troppa attenzione alle clausole di invarianza finanziaria, che vengono ripetute nel testo, quasi come fossero un *mantra*: ogni tanto sembra quasi una *excusatio non petita*, ma sarà poi compito del Governo riuscire a far quadrare i conti, da questo punto di vista. È importante anche l'attenzione che il testo riserva sia al sistema tavolare, nelle Regioni in cui esso è presente, sia alle specificità delle Regioni a statuto speciale, per cui si prevede un rinvio alla normativa di attuazione, che è già presente e che dovrà essere integrata e modificata, in seguito all'approvazione del testo in esame, per tener conto delle modifiche apportate. Certo, il quadro attuale è preoccupante e la senatrice Stefani lo ha descritto in maniera molto dettagliata e puntuale, ma proprio per questo è necessario fare un passo in avanti, sapendo benissimo che è soltanto un passo all'interno di un processo più ampio. È indispensabile farlo perché l'alternativa è restare nella situazione che la senatrice Stefani ha testé descritto bene e anche impietosamente, sapendo che si tratta di un tassello all'interno di un mosaico assai più complesso di riforma del sistema giudiziario

La magistratura onoraria assolve quindi a un compito fondamentale e vitale per il buon funzionamento della giustizia, ma nello stesso tempo gode di un trattamento giuridico e ordinamentale inadeguato rispetto all'importanza della funzione svolta. È quindi necessario garantire alla magistratura onoraria alcune garanzie giuslavoristiche al fine di poter assicurare professionalità, indipendenza e imparzialità,

di alcuna forma di tutela assistenziale e previdenziale, non maturano il diritto alla pensione, non godono di tutela alcuna per la salute, la gravidanza, la famiglia, gli infortuni sul lavoro e non è nemmeno previsto un trattamento di fine rapporto. La delega prevede infatti di individuare e regolare un regime previdenziale e assistenziale compatibile con la natura onoraria dell'incarico, ma - si specifica - senza oneri per la finanza pubblica, prevedendo l'acquisizione delle risorse necessarie mediante misure incidenti sull'indennità. È evidente che l'inciso «senza oneri per la finanza pubblica» andrà a garantire alcun diritto o, al massimo, garantire qualche diritto dimezzato e certamente ciò inciderà anche sulla retribuzione. In particolare, i diritti costituzionali alla salute e alla maternità risulterebbero lesi dalla previsione della dispensa per qualsiasi impedimento che si protragga per sei mesi, come previsto dall'articolo 2, comma 10, lettera *a)*, del presente disegno di legge delega. Anche per quanto riguarda i compensi, il testo, prevedendo che l'indennità dei giudici di pace deve essere inferiore a quella prevista per l'esercizio di funzioni giurisdizionali, evita ogni riferimento quantitativo e, inoltre, collega la corresponsione della parte variabile al grado di raggiungimento degli obiettivi e comunque rimette la valutazione di tali obiettivi al parere discrezionale del presidente del tribunale.

e non ricollegato a parametri variabili determinati dal presidente del tribunale. Queste disposizioni, peraltro, contrastano con le recenti posizioni prese dalle più alte istituzioni europee con l'apertura della procedura di infrazione avviata dalla Commissione europea nei confronti dello Stato italiano che, proprio a seguito di denuncia di un magistrato onorario italiano, ha sollevato - come sappiamo - la questione di compatibilità delle condizioni di lavoro

Tra l'altro, i magistrati in servizio da oltre dodici anni avrebbero anche raggiunto il diritto alla stabilizzazione sulla base della direttiva comunitaria sul lavoro a tempo determinato. Anche la previsione di un numero limitato di mandati, confermata dalla delega, non può essere ammissibile per i magistrati in regime transitorio, che svolgono un delicato compito giurisdizionale e che a causa del progressivo aumento della competenza non riescono a svolgere altra attività professionale.

e che, con la previsione di un numero limitato di mandati, si troverebbe improvvisamente, all'età di circa sessant'anni, tagliata fuori dal mondo del lavoro. Si sottolinea che la maggior parte dei giudici di pace attualmente in servizio ha dovuto dismettere ogni altra attività lavorativa, per cui la riforma creerebbe probabilmente ulteriori esodati, magistrati che non avranno né retribuzione né previdenza. Quindi, non potrà prevedersi un periodo di permanenza nelle funzioni inferiore a venti anni, a pena di non maturare nemmeno i requisiti minimi di pensionamento. Per questo pensiamo che si potrebbe prevedere, già nella delega, una graduatoria ad esaurimento solo per coloro che ne facciano richiesta e che svolgano le funzioni di magistrato onorario da almeno dieci anni, e comunque a decorrere solo dal momento in cui divenga attuativo la presente delega.

necessaria ad un efficiente funzionamento degli uffici di giustizia, viene visto in maniera critica da molti soggetti interessati. Siccome pensiamo che stiamo ancora una volta approvando una riforma monca, che non tutela la magistratura onoraria,

farò un'esposizione brevissima e molto sintetica, per tratti davvero salienti, della posizione del nostro Gruppo, che - anticipo - voterà a favore del provvedimento. Le ragioni per le quali siamo favorevoli a questo disegno di legge, che delega il Governo a provvedere sul tema variegato della magistratura onoraria, sono presto dette. la funzione temporanea della magistratura onoraria ha provocato, con il reiterarsi di incarichi conferiti e ancora prorogati, una definizione che è stata appropriatamente indicata con un ossimoro: la «precaria stabilizzazione». si pone un quadro di insieme molto più coerente e ben articolato. Intanto, viene definito uno statuto unico della magistratura onoraria, con una disciplina omogenea nelle sue varie articolazioni (giudice di pace, giudice onorario, vice procuratore onorario) per quanto riguarda l'accesso, la durata, la formazione, il sistema disciplinare e anche le garanzie del principio di indipendenza, che comunque devono presiedere a qualsiasi forma di giurisdizione, sia essa ordinaria od onoraria. Viene anche superato quel concetto deteriore che attribuiva alla magistratura onoraria il mero compito di supplenza in sostituzione del giudice ordinario

È anche stata appropriatamente introdotta una normativa che attiene al doppio regime che distingue la posizione dei magistrati onorari in servizio da quelli di nuova assunzione. Nell'impiego della magistratura onoraria nelle varie articolazioni del processo viene fatta chiarezza con una normativa puntuale. Vengo ora ad un'ultima osservazione relativa ai compensi

segue: «prevedere che l'indennità debba essere corrisposta con modalità idonee ad assicurare la previa verifica, da parte del presidente del tribunale per i giudici onorari di pace e da parte del procuratore della Repubblica per i vice procuratori onorari, del raggiungimento degli obiettivi stabiliti». Viene quindi posto in funzione un doppio binario di attribuzione di compensi:

ed è bene precisarlo e questa è l'ultima osservazione che faccio - non viene indicato un criterio meramente quantitativo, una sorta di cottimo, per così dire, per premiare l'efficienza

Queste sono le mie osservazioni. Al di là di qualche critica, che non rievoco ma che può essere condivisa da parte di chi è intervenuto contestando qua e là alcuni punti della norma, nel complesso e rispetto alla situazione preesistente di confusione e di

Signor Presidente, anticipo subito che il Gruppo del Movimento 5 Stelle voterà contro questo disegno di legge. Sarà un no nel merito,

Certo, è una disciplina che finalmente detta regole che mancavano da anni e che dà un orizzonte temporale e una sistemazione più o meno organica alla materia - ed quello che ci si aspettava - però le regole proposte in questo disegno di legge non ci convincono a tal punto da votare a favore. Nonostante il nostro voto negativo di oggi, ovviamente, qualora nel successivo passaggio parlamentare

Intanto notiamo che, a testo vigente, così come licenziato dopo la fase emendativa, è previsto un aumento della dotazione organica un dimezzamento del lavoro. C'è una sostanziale riduzione dei compensi, dovuta all'impiego intensivo dei tirocinanti nell'ufficio per il processo, che imporrà a tutti i magistrati onorari di cercare un'attività di lavoro complementare. Dalla scelta operata prima, tra tempo pieno e semipieno, si passerà verosimilmente per legge all'impiego semipieno di tutti i magistrati onorari. Quindi, quale vantaggio ci potrà essere per la giustizia se il magistrato dovrà dividersi su più fronti, dove da un lato c'è il lavoro che dovrà dare il sostentamento per la vita e, dall'altro, c'è la prospettiva lavorativa di un incarico onorario con una data di scadenza? Questa previsione comporterà una dispersione delle professionalità dei magistrati più esperti prima ancora che essi decadano per fine mandato, perché si imporrà loro di cercare altre fonti di reddito, condizionando in modo negativo l'esercizio delle funzioni giurisdizionali con ogni evidenza anche una problematica conflittuale nello svolgere una professione così delicata come la funzione giurisdizionale insieme alla libera professione o ad altri rapporti di lavoro dipendente. A tal proposito avevamo proposto consapevoli che la sua portata era molto incisiva e avrebbe meritato un maggior tempo di riflessione e di dibattito tra i Gruppi parlamentari, ma non c'è stata la possibilità. Quell'emendamento, qualora fosse stato approvato (ma non dubito che sarà riproposto dai nostri colleghi alla Camera),

per un regime di incompatibilità con altre professioni. Infatti, il problema tipico - diciamocelo - è quello di chi fa il magistrato onorario ed è anche avvocato ed è autorizzato a esercitare la libera professione al di fuori del distretto in cui svolge funzioni giurisdizionali. Questo non comporta un conflitto diretto, ma è pur sempre una distorsione del principio, al quale dovremmo attenerci, del magistrato terzo, libero e indipendente. Se avessimo potuto dare la facoltà di optare per un regime di incompatibilità, accompagnando «su richiesta», fino al settantesimo anno di età, questi magistrati che avrebbero voluto dedicare tutte le proprie energie a

di astensione obbligatoria per maternità, che dura almeno cinque mesi, a sopravvivere senza alcun tipo di retribuzione. Festeggiare allora

Camera, per garantire continuità contributiva almeno per coloro che opterebbero per un regime di incompatibilità. Queste persone direbbero: «Faccio il magistrato onorario, faccio solo questo non faccio altro; cerco anche di farlo bene e sono sottoposto a tutti i giudizi di qualità, ma che mi siano garantite almeno quelle condizioni minime, come, ad esempio, la continuità contributiva»; noi l'avevamo proposta,

del Partito Democratico esposto dall'attuale Ministro della giustizia, che all'epoca era il responsabile del settore giustizia del Partito Democratico, in un incontro di Magistratura democratica, relativamente alla magistratura onoraria

faceva infatti espresso riferimento ad una disciplina transitoria che avrebbe dovuto garantire la conferma dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio alla data di entrata in vigore della legge per mandati ulteriori quadriennali fino al compimento del settantesimo anno di età.

che noi sosteniamo. Si prevede poi che i magistrati onorari debbano adottare provvedimenti in conformità alle direttive del magistrato professionale. di un pericoloso principio che, al di là di una ragionevole attività di coordinamento interpretativo, giurisprudenziale o di prassi giurisprudenziale in ambito distrettuale o di tribunale, implica il rischio di una sottoposizione del magistrato onorario alle direttive

prestavano, al di là della formale onorarietà della funzione, si indirizzava secondo le direttive di un superiore e questo potrebbe

che un provvedimento di archiviazione o comunque assolutorio. Questo non tranquillizza il cittadino, che dovrebbe avere il diritto di approcciarsi alla giustizia sapendo di trovarsi dinanzi un giudice che, togato od onorario, è nella condizione di essere veramente libero, indipendente e terzo, senza i condizionamenti impliciti che potrebbe avere sapendo che la propria retribuzione dipende

gioia, anzi, con grande rammarico il Gruppo di Forza Italia voterà contro questo provvedimento, ancorché il nostro Gruppo sia stato quello che sin dal 2011 una seria modifica dell'ordinamento dei giudici onorari. Perché voteremo contro? Perché questo provvedimento, ancorché abbia ricevuto, grazie anche alla nostra insistenza, alcune alcune significative modifiche, in particolare sui quattro quadrienni di permanenza in servizio per quelli che oggi sono in servizio, servizio, risente, per alcuni aspetti, di una idea sbagliata. Tale idea vuole i giudici onorari come non legittimati a esercitare la giurisdizione. Un'idea che traspare dal tessuto di questa legge delega, che dimostra, a più riprese e in più punti, la mancanza di fiducia di apprezzamento del lavoro svolto dai giudici onorari, e ciò in contrasto con la nostra Costituzione. La Costituzione italiana, al comma 2 dell'articolo 106, espressamente dice: «La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva,

Noi abbiamo scelto, con la Costituzione, il modello del giudice incasellato con il concorso in un sistema burocratico. vince il concorso e fa il giudice. In altri sistemi, invece, il giudice ripete la propria legittimazione ad esercitare la giurisdizione dall'elezione popolare. Il giudice selezionato per concorso ripete la propria legittimazione dalla professionalità e dall'aggiornamento continuo rispetto al momento iniziale del concorso. Aver previsto per i giudici onorari la possibilità della elezione vuol dire quindi che il giudice onorario aveva una tale legittimazione da essere previsto come giudice singolo, con la sostituzione delle funzioni del giudice di carriera che svolge quelle funzioni da solo. Invece, noi ci siamo ritrovati una legge delega di completa sfiducia,

Che questo sia un ulteriore errore lo dimostra il fatto che avete ricopiato la condizione da me indicata, che legittimava l'attribuzione di procedimenti singoli

che introduceva i GOT in tribunale esclusivamente quale supplenza del giudice mancante e non con l'attribuzione di una competenza propria. propria. Rispetto a questa soluzione abbiamo sottolineato alcune incongruenze, mentre abbiamo apprezzato altri aspetti. Ci siamo battuti sin dall'inizio,

mi sono permesso di dire quantomeno che siano quelli attualmente in vigore. Ma la Commissione bilancio dice che c'è l'apertura verso l'alto, non c'è un limite. Ma verso l'alto non c'è un limite: nella legge che state approvando non solo non c'è un limite, ma addirittura nella normativa sull'invarianza della spesa introducete un criterio un criterio con la consapevolezza che quei decreti legislativi potranno non avere la copertura. Quindi sarete costretti a dire che i decreti non entreranno in vigore e il Governo dovrà reperire i fondi per la copertura. avete sfiducia nei confronti di questi soggetti, che invece avrebbero avuto necessità, proprio per il lavoro che svolgono, un apprezzamento fondamentale. Vedete, la giurisdizione è unica e mi dispiace che il Capigruppo del PD nella Commissione giustizia, il senatore Lumia, probabilmente non attenzione, così come non abbiamo attenzione tutti noi, con responsabilità del mio Gruppo e di tutti i Gruppi. Quando si tratta dei diritti dei cittadini vi è disattenzione in quest'Aula,

Com'è possibile accettare che vi sia una non considerazione della giurisdizione? Sono principi fondamentali

che non era possibile, per il potere di condizionamento che aveva, un parere dell'Ordine degli avvocati per i magistrati ordinari in occasione della valutazione di professionalità o delle promozioni. Come potete oggi inserire una cosa del genere per quanto riguarda la conferma? Vi rendete conto che questo significa condizionare il giudice onorario alla conferma dell'avvocato famoso, influente nel proprio consiglio dell'ordine, che potrebbe dare indicazioni di non conferma? Quale utilità avete nel voler introdurre per forza una norma generica sulla previdenza e sull'assistenza quando non avete introdotto nemmeno una norma sulla gravidanza? Com'è possibile che voi diciate che dovremmo fare una previdenza generica con le indennità senza dirci nulla dei giudici onorari e quando fate una costruzione che ci lascia presupporre forse una diminuzione dei compensi? Manca del tutto l'attenzione;

signor rappresentante del Governo? Ci vuol dire quando saremo in grado di poter assicurare e programmare l'impegno di attività della giustizia? Sappiamo tutti quello che danno. Qual è il programma, come organizzarsi? Manca un mese e mezzo. Come possono organizzarsi i giudici onorari, i presidenti di tribunale e i capi degli uffici che devono organizzare il lavoro? Non avete dato nulla, nemmeno per la proroga. Concludo

insieme; altre, però denunciano - da un lato - una non considerazione del lavoro svolto dalla magistratura onoraria e - dall'altro - una genericità che lascia perplessi non ci consente di esprimere una valutazione effettiva di qual è l'intendimento del Governo. Avremmo avuto la necessità di garantire con precisione quanto tempo può durare l'applicazione all'ufficio per il processo di uno che ha superato il primo biennio quali sono i termini che bisogna introdurre per il tirocinio. E invece, non c'è nulla. Per questa ragione, signor Presidente, nonostante gli aspetti positivi, per riaffermare la forte valenza della magistratura onoraria per una corretta amministrazione della giustizia nel nostro Paese, voteremo contro.

una riforma attesa da tanti e tanti anni. Molti Governi si sono succeduti, ma nessuno è riuscito a proporre una riforma condivisa dal Parlamento. Ricordo a tutti i senatori che, oltre alla legge delega del Governo, erano in campo ben sei disegni di legge da parte dei vari Gruppi parlamentari, compreso naturalmente quello del Partito Democratico. Ricordo ai colleghi che i giudici onorari attendono da tanti e tanti anni una riforma: 1998 (sono passati ben diciotto anni), 2008 (sono passati ben otto anni), 2009 (sono passati ben sette anni). Ecco perché anche questa riforma qualifica e caratterizza il lavoro della maggioranza, del Governo e debbo dire anche del Senato. Così è stato in Commissione giustizia, dove c'è stata un'ampia condivisione intorno al testo che il relatore ha presentato qui in Aula. Ma poi, siccome in Aula spesso prevalgono ragioni politiche, che sono spesso - ahimè - estranee al merito, ecco la disarticolazione e il voto contrario di Gruppi dell'opposizione. Colleghi, ricordo a tutti che finalmente diamo in esercizio alcune norme previste dalla nostra Costituzione agli articoli 102 e 106. Questa riforma organica finalmente sottopone la magistratura

Noi, cari colleghi, ringraziamo la magistratura onoraria, che svolge una funzione importante nel nostro sistema e ha un carico importante. Ma condividiamo, con la parte più avanzata della loro rappresentanza, la necessità di fare un bel salto di qualità, bel salto di qualità, in grado di dare efficienza al loro ruolo e dignità alla loro funzione, integrandola meglio con la magistratura professionale e responsabilizzandola all'interno di obiettivi di cambiamento e di miglioramento dell'offerta del servizio giustizia.

prevede adesso l'inserimento nell'ufficio del giudice di pace anche degli attuali giudici onorari di tribunale, superando la distinzione tra le due figure, che vengono ridenominate giudici onorari di pace. previsto l'inserimento nella magistratura requirente onoraria, in un'articolazione denominata ufficio dei vice procuratori onorari, all'interno dell'ufficio della procura della Repubblica presso il tribunale ordinario.

salvi gli effetti della riabilitazione. Sono state date delle indicazioni sulle modalità di accesso alla magistratura onoraria e previsti titoli preferenziali per la nomina a magistrato onorario a favore di coloro che hanno esercitato funzioni giudiziarie a titolo onorario, avvocati, notai

istruire e valutare le domande, formulare, all'esito del tirocinio gratuito da svolgersi presso un magistrato professionale affidatario, un giudizio di idoneità e proporre una graduatoria degli idonei per la nomina a magistrati ordinari.

previsione che, dopo il primo incarico quadriennale, la funzione di giudice onorario di pace possa essere confermata solo per un altro quadriennio e, quindi, la durata complessiva dell'incarico non possa superare complessivamente gli otto anni.

Abbiamo anche previsto un regime transitorio importante per i magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi,

da migliorare, come spesso è stato detto in Commissione e ribadito dal relatore nella relazione illustrativa dell'importante disegno di legge

Il fatto che si stia disciplinando la cosiddetta magistratura onoraria non ci deve indurre a pensare che i suoi magistrati siano di serie B, perché gli effetti delle sentenze da essi emesse da essi emesse non sono di rango inferiore. Esse attengono a specifiche casistiche che non hanno particolare rilevanza sotto il profilo delle libertà dei cittadini, ma colpiscono nel vivo interessi e questioni che non possono essere ritenuti di secondo ordine. Ricordo a me stesso che l'istituto del magistrato onorario è stato un pannicello caldo adottato qualche tempo fa di fronte all'impotenza, alla farraginosità e alle lungaggini la magistratura cosiddetta ufficiale aveva e tuttora fa registrare rispetto alla velocità dei processi e, quindi, alla certezza del diritto

un aspetto che riguarda la giustizia in quanto tale, e non una giustizia di serie B. sia possibile immaginare una retribuzione a questo magistrato, per quanto onorario, diversificata rispetto al tipo di sentenza che emette. Se emette una sentenza di archiviazione, mi pare si tratti di una decina di euro. Se, invece, rinvia a giudizio, la remunerazione aumenta.

Cucca è stato più volte sollecitato a rispondere, ma io mi domando: non è questa un'ingerenza del legislatore? Non è questo un poco ortodosso indirizzo che il legislatore dà

un'ulteriore invadenza della legislazione verso determinazioni che il magistrato dovrebbe assumere in piena autonomia e senza altri pregiudizi o interessi? Credo che stiamo andando, ancora una volta, oltre quelli che dovrebbero essere il ruolo e la funzione dello Stato. Il senatore Lumia ci ha ricordato con grande eleganza che questo fa parte della riforma della giustizia e che prima le riforme si facevano *ad personam*. Lumia immagina che le leggi si debbano fare *contra personam* perché, se prima si facevano a favore delle persone, adesso le facciamo contro le persone.

ai Gruppi, alle ore 12 sarà ricordato il settantesimo anniversario del riconoscimento del diritto di voto alle donne in Italia. Sospendo pertanto la seduta fino alle ore 12.

era il 10 marzo del 1946, settant'anni fa, il giorno del primo voto delle donne italiane. Per decidere se riconoscere o no il voto alle donne, la strada è stata molto lunga, sono stati fatti tanti atti e tanti approfondimenti. Pensate, fu fatta perfino una sorta di sondaggio all'inizio del Novecento,

La prima è quella della docente, professoressa universitaria dell'università di Pavia, Rina Monti. Alla prima domanda («Si deve riconoscere il diritto di voto (...) alle donne?»), lei rispose in generale, sì, si può fare, «perché ogni diritto deve essere conquistato da chi ne sente la mancanza. Nessuna concessione è proficua a chi non ne conosca il valore». Alla seconda domanda (estenderebbe il voto alle donne oggi,) la professoressa Rina Monti rispose no (parliamo del 1905), argomentando: «perché il voto alle donne oggi in Italia segnerebbe l'avvento di una reazione politica, amministrativa e intellettuale, quale non si è mai vista». E prosegue: sono ancora troppo ignare della vita pubblica, troppo lontane da ogni educazione positiva, e perciò schiave del pregiudizio religioso, che le rende docili istrumenti dei preti, depositarie di tutte le idee antiquate, di tutti gli errori secolari, di tutto il misoneismo antiscientifico. Prima di dare il voto alle donne è necessario rendere viva e moderna la loro educazione, distruggere i loro pregiudizi atavici, dare loro una personalità indipendente. È tutto un lungo lavoro che resta da fare». Era il 1905. Ma nello stesso sondaggio e nella stessa indagine conoscitiva venne ascoltata la professoressa Maria Montessori, che tutti noi ancora oggi ricordiamo. E lei, invece, rispose fermamente di sì: bisogna dare il voto alle donne subito, oggi,

c'è tanto numero di lavoratrici fra operaie, maestre, impiegate nelle pubbliche amministrazioni, anch'esse portano un serio contributo al lavoro sociale: mentre non hanno i diritti dell'uomo e i suoi compensi al proprio lavoro. Per raggiungere l'opera di giustizia sul lavoro della donna è necessaria la solidarietà e la difesa parlamentare». Attenti, colleghi, era il 1905 e la Montessori diceva: non si troveranno deputati che per la solidarietà e la difesa della donna dedichino la loro esistenza di uomini politici - come sarebbe necessario - se le donne non potranno dare il loro voto, cioè farli eleggere deputati». Ecco, era il 1905 1905 e da quell'indagine conoscitiva si arrivò al 1946. Quelle del 10 marzo 1946 erano le elezioni amministrative, le prime elezioni amministrative dopo il fascismo, che rinnovavano 436 Comuni. Tutte le italiane che avevano compiuto ventuno anni votarono per la prima volta. Erano le prime elezioni libere dal fascismo e quello stesso giorno fu molto importante, perché alle donne italiane alle donne italiane venne riconosciuto, con un decreto, anche il diritto all'elettorato passivo. Proprio con quelle elezioni, un grande numero di donne - pensate, solo ventuno, ma per quell'epoca tantissime su oltre 500 seggi - vennero elette alla Costituente; un gruppo di donne a cui va il mio e il nostro pensiero; donne che hanno fatto la storia dell'Italia e della nostra democrazia. Il 2 giugno dello stesso anno le donne furono chiamate anche al voto referendario per scegliere tra la monarchia e la Repubblica. ho trovato una bellissima testimonianza, richiamata dalla presidente Fedeli qualche giorno fa, di una giornalista, Anna Garofalo, che così racconta quel giorno:

quel simbolo, quel segno, una crocetta accanto a quel nome. Stringiamo le schede come biglietti d'amore.

questo accadeva in quegli anni in cui le donne si apprestavano ad ottenere il loro primo diritto di voto. noi abbiamo, prepotente, ancora una questione da affrontare che è quella della rappresentanza di genere, che si è spostata sull'avanzamento della democrazia paritaria. In questo Senato, grazie al lavoro di tutte noi, abbiamo, negli ultimi mesi, ottenuto risultati importanti. Penso alla modifica delle regole per le elezioni dei membri del Parlamento europeo. Penso alla nuova legge elettorale che prevede la doppia preferenza di genere, che già abbiamo testato testato e sperimentato in alcuni Comuni, e alla norma antidiscriminatoria che vieta di superare il 60 per cento di candidati dello stesso sesso tra i capilista. La vera conquista per la quale dobbiamo ancora tutte lavorare è proprio questa: ottenere la rappresentanza paritaria delle donne in quei luoghi dove si svolgono i processi decisionali. Anche da questo dipenderà la qualità futura della nostra democrazia. A tale proposito, però, è necessario un grande sforzo educativo e culturale. È bene che nelle nostre scuole sia fatto un grande lavoro di studio e di approfondimento sul contributo delle donne in tutto il percorso repubblicano, non solo per ossequiare l'articolo 51 della Costituzione. Riflettiamo insieme, colleghe, noi per prime, su quanto sia scontato per le nostre figlie e nipoti il diritto di rappresentanza di genere. Le nostre ragazze vanno a votare, o peggio scelgono di non andare a votare, considerando questo un diritto acquisito, un diritto scontato, un diritto dovuto. Per loro la memoria è ancora troppo corta, soprattutto - penso - per causa nostra. Ecco, è in questo grave rischio di irrilevanza che io vedo ancora grossi vuoti culturali. Abbiamo ancora da raggiungere molti obiettivi e moltissimi ne raggiungeremo a breve. Penso alla piena attuazione della attuazione della Convenzione di Istanbul, uno dei primi atti votati in questo Senato, appena ci siamo insediati, che ha l'obiettivo di stroncare l'orribile piaga della violenza contro le donne. Ricordo che c'è ancora molta strada da fare, soprattutto in termini educativi. Dobbiamo rendere la maternità davvero una libera scelta, lottando contro le dimissioni in bianco e dando concretezza all'estensione dei congedi di maternità e paternità. Tutte insieme dobbiamo ancora fermare le penalizzazioni esistenti sui luoghi di lavoro - pensate alle discriminazioni retributive - e infine ottemperare pienamente a quegli obblighi costituzionali previsti dagli articoli 3 e 51, per ottenere un maggiore equilibrio tra uomini e donne nelle Assemblee elettive. Vi ricordo che, nella civile Italia e nella moderna lotta per la rappresentanza paritaria, esistono ancora Regioni con una sola eletta e una Regione, la Basilicata, con un Consiglio regionale di soli uomini. Signor Presidente, oggi ricorre il settantesimo anniversario del voto alle donne che, nel periodo del fascismo, fu inopportunamente impedito. In quel periodo di limitazioni di libertà le donne venivano considerate il pilastro del nucleo familiare, ma nulla di più. Nel 1946, finalmente, tornata la democrazia, le donne poterono diventare protagoniste della società, dando

che ancora purtroppo scontano alcuni pregiudizi e un *gap* in determinati ruoli, ma anche disparità rispetto agli uomini nelle retribuzioni e nei livelli delle pensioni. Ma questo divario in Italia si va colmando e le donne acquistano, sempre più, nuovi ruoli da protagoniste nella scuola e nel lavoro. Siamo storicamente a un livello più avanzato nella funzione della donna nella società. Oggi le donne siedono in Parlamento, nelle istituzioni più autorevoli e nei consigli di amministrazione delle società che fanno crescere il nostro Paese. Il nostro pensiero, in questi giorni, va certamente alle donne di quei territori del mondo che, in nome di interpretazioni delle leggi islamiche date dagli uomini, subiscono brutali limitazioni, e non solo al diritto di voto, ma anche alla loro stessa libertà. Ma non dimentichiamoci nemmeno che, mentre noi stiamo parlando, in qualche parte d'Italia o del mondo, una donna sta subendo una violenza. Così come non scordiamo l'aberrante fenomeno del femminicidio quasi come fatto quotidiano. Dobbiamo dare dignità alla donna, aiutarla a stare a testa alta, in ogni ambito e in ogni ruolo che ricopre. Il nostro lavoro di legislatori è chiudere definitivamente ogni divario tra uomo e donna in Italia e operare affinché nei consessi internazionali prevalga la determinazione a restituire libertà alle donne, in ogni parte del mondo. Il nostro obiettivo guarda a quelle grandi democrazie occidentali dove il ruolo della donna che contrassegna i livelli apicali della società e persegue il progresso in campo economico e scientifico. E in questo senso il nostro ringraziamento va a tutte quelle donne italiane che, nei consessi internazionali ricoprono, ruoli di stimolo all'innovazione e alla crescita del benessere nel pianeta. Ma non ci dimentichiamo che ogni obiettivo legittimo di carriera può e deve essere coniugato con il ruolo principale di ogni donna, quello di essere madre, al centro della famiglia, ma con più diritti e più aspettative rispetto al passato. Mi auguro, quindi, che la società contemporanea evolva sempre più nella direzione di garantire alle donne maggiore presenza attiva e più diritti.

onorevoli senatori, c'è un giorno della storia sempre poco rimarcato: un giorno di settant'anni fa, in cui le donne italiane per la prima volta abbandonarono per qualche ora il focolare domestico e si misero in fila davanti ai seggi in una Nazione ancora semidistrutta dalla guerra. Quel giorno non fu, come in tanti credono, il 2 giugno 1946, quando si votò per scegliere tra monarchia e Repubblica ed eleggere l'Assemblea costituente. Quasi tre mesi prima, il 10 marzo di quello stesso anno, si tenne infatti la prima tornata di elezioni amministrative che avrebbero portato ai primi sindaci eletti dopo il Ventennio. E a votare sarebbero stati i cittadini di entrambi i sessi: una conquista arrivata dopo anni di battaglie e molto più tardi rispetto ad altre donne europee e statunitensi. Le donne e il diritto di voto: è un fatto che sembra scontato, ma fino alla metà del secolo scorso non lo era affatto. Scorrendo la classifica mondiale dei Paesi che per primi hanno approvato il suffragio femminile, in testa c'è la Nuova Zelanda nel 1893, seguita dall'Australia e dai Paesi scandinavi ai primi del Novecento, poi dalla Russia, con la Rivoluzione d'ottobre, la Gran Bretagna e la Germania dopo la Prima guerra mondiale e gli Stati Uniti nel 1920. L'Italia approva il suffragio femminile solo alla fine dell'ultima guerra, solo dopo un percorso lungo e difficoltoso, iniziato nel lontano 1877, quando Anna Maria Mozzoni, considerata la pioniera del nostro femminismo, presenta al Parlamento la prima petizione a favore del voto femminile. Da allora ci sono voluti altri settant'anni prima che le donne italiane potessero cominciare ad esprimere la propria opinione politica attraverso il voto. L'affluenza delle donne ai seggi elettorali fu altissima e la partecipazione emotiva intensa. In quelle prime domeniche di democrazia, dopo anni di dittatura e guerra, oltre l'89 per cento delle donne aventi diritto si recò alle urne, mentre nei diversi consigli comunali furono elette 2.000 candidate. Le votazioni si svolsero in cinque tornate primaverili con l'elezione di quasi 6.000 amministrazioni e il coinvolgimento del 71 per cento della popolazione italiana. Si votò dal 10 marzo, ogni domenica, fino al 7 aprile, mentre altri 1.400 comuni furono rinnovati in autunno, con altre otto tornate tra ottobre e novembre. Una prima presenza femminile si ebbe nella Consulta nazionale. L'assemblea non elettiva, composta dai esponenti dei partiti del Comitato di liberazione nazionale, funse da Parlamento tra il 1945 e il 2 giugno 1946 e vide la nomina di 13 donne su 460 membri. I partiti stessi, almeno quelli che erano emersi più forti dalla Guerra di liberazione, avevano ormai intuito che era arrivata l'ora del voto. La Democrazia Cristiana e il Partito Comunista italiano erano consapevoli che si stava per costruire un nuovo sistema di democrazia di massa e sarebbe stato anacronistico edificarlo senza le donne. Sulla questione del voto, fondamentali furono poi le parole di papa Pio XII che diede in un certo senso la sua benedizione, dopo che per lungo tempo la Chiesa di Roma aveva visto con terrore la possibilità che le donne andassero a votare. La conquista del diritto di voto è stata sentita dalla donna come il primo fondamentale passo per il suo processo di emancipazione, che è riconoscimento di pari diritti con l'uomo e insieme della sua identità. Il diritto di voto non è stato sentito solo come il diritto di scegliere i propri rappresentanti politici e di potere essere elette, ma come l'abbattimento di una serie di norme che vedevano la donna subalterna all'uomo, a partire dalla mancanza di autonomia economica. Il diritto al voto ha quindi aperto la strada alla conquista di una società più democratica. Nell'ambito sociale, inoltre, vanno sottolineati molti cambiamenti che hanno riguardato le donne e la loro partecipazione al mercato del lavoro, alla vita familiare e ai gradi di istruzione. È la stessa Corte costituzionale, nel 1960, a dichiarare illegittima la norma che escludeva le donne da una vasta categoria di uffici pubblici. Negli anni successivi, il legislatore con una serie di provvedimenti e di leggi ha consentito ha consentito una sempre maggiore parità sostanziale, migliorando notevolmente la situazione in molti settori strategici per il nostro Paese, come quelli sociale, lavorativo ed educativo. Tuttavia, alcuni dati ufficiali della presenza femminile nelle istituzioni mettono in luce che c'è ancora molta strada da percorrere. Purtroppo, ancora oggi, secondo dati ISTAT del 2013, tra gli amministratori comunali in carica, il 78,7 per cento sono uomini e solo il 21,3 donne; solo l'11,7 per cento sono sindaci donne e nell'attuale Parlamento italiano, tra l'altro con la maggior presenza femminile nella storia repubblicana, le donne costituiscono solo il 30 per cento. Molta strada rimane ancora da fare. Anche l'OCSE, con uno studio pubblicato proprio in occasione della giornata delle donne, ha ricordato come la riduzione della partecipazione femminile alla forza lavoro e alla produttività totale, che deriva dal mancato completamento della parità di genere nella società e nel mondo del lavoro, abbia un impatto sostanziale sull'economia globale, con un costo in termini diretti di circa 12.000 miliardi di dollari, pari al 16 per cento del prodotto interno lordo mondiale. L'organismo internazionale esorta quindi le singole nazioni ad eliminare la discriminazione verso le donne e a promuovere le pari opportunità, definendole sia scelte economicamente intelligenti, sia leve importanti per una crescita sostenibile ed inclusiva. Esiste, quindi, ancora uno scarto tra la parità formale, pronunciata e celebrata in ogni occasione, e la parità sostanziale tra uomini e donne, quest'ultima molto più difficile da realizzare. Ed è in questo senso che ancora bisogna lavorare: devono lavorare le istituzioni, si deve impegnare la politica, deve agire anche la società civile. Il settore privato deve sostenere il pubblico nell'erogazione dei servizi. Bisogna diffondere una cultura della parità in tutti i livelli della società e bisogna spiegare alle bambine di quali conquiste oggi possono beneficiare. E devono essere anche e soprattutto le donne a fare questo, esattamente come devono continuare nell'impegno per la propria affermazione e realizzazione, senza quote e senza riserve, per il riconoscimento del loro corretto ruolo nella società, con dignità e coraggio. Per concludere, vorrei citare le ultime conquiste che la sensibilità di questo Parlamento ha ottenuto in tema di parità di genere nella rappresentanza politica. In particolare, con la riforma costituzionale sono state inserite nella Carta alcune disposizioni in tema di parità di genere nella composizione delle nuove Camere, così come nella composizione dei Consigli regionali. E, ancora, ricordo la nuova legge elettorale per la Camera dei deputati con le norme in favore della rappresentanza di genere, sia nella successione alternata nelle liste, sia nel numero dei capilista.

gentili colleghi e gentili colleghe, è bello celebrare le donne ma, nel momento in cui le si celebra, si è ancora lontani dalla parità. Quindi, mi mette molta tristezza, anche oggi, dover celebrare il voto della donne quando siamo ormai oltre, quando Non voglio fare un riassunto di tutte le conquiste per le donne, già fatto dalle mie colleghe. Il diritto di voto mi sembra il minimo. In questi settant'anni, però, oltre al diritto di voto si è fatto molto poco perché, come emerge da una relazione dell'organizzazione non governativa Oxfam Italia, quello che la storia non ci insegna riguardo al diritto delle donne è il vero costo della disuguaglianza e dell'austerità in Europa. infatti parlare di quote rosa, di quante donne siedono in Parlamento, di quante sono presenti nelle istituzioni e di quante lavorano, ma pochi si soffermano a vedere cosa sia la vita delle donne nella società. La vita delle donne nella società, purtroppo, è quella di sostituire uno Stato sociale che non esiste più. Al di là di quanto dicono poi le celebrazioni di questo Parlamento, dove siamo molto tutelate e privilegiate (sia uomini che donne), la vita delle donne nelle città è molto diversa.

quando si hanno dei genitori anziani, per i quali non c'è assistenza; quando non c'è una sanità che ti sorregge; quando hai delle amiche che subiscono violenza e ti dicono che non sanno dove andare, perché nessuno le aiuta, perché non esistono più i consultori e non esiste più assistenza. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Questa è la vera libertà delle donne. Possiamo anche farle votare, ma non ne hanno neanche più voglia, perché nessuno le aiuta. Inutile invocare le quote rose e la riforma costituzionale per le donne. La riforma costituzionale è per dare ancora più potere a chi lo detiene e ha delegato le donne all'ultimo posto. Vi dovreste vergognare a invocare la riforma costituzionale per la tutela delle donne!

voglio parlarvi di tale questione, perché è facile dire che si prevedono le quote rosa quando poi andiamo in Europa e non battiamo i pugni sul tavolo per dare sostegno alle famiglie in difficoltà. Anche perché è nelle famiglie che lavorano le donne. che lavorano le donne. Il rapporto Oxfam Italia, «Il vero costo della disuguaglianza e dell'austerità in Europa», pubblicato nel settembre 2013, nel solo 2011, 120 milioni di persone nell'Unione europea hanno dovuto affrontare la prospettiva di vivere in povertà. Oxfam calcola che questo numero potrebbe crescere di almeno 15 milioni, come risultato delle prolungate misure di austerità. Tra i nuovi poveri si sa già che le donne saranno quelle maggiormente colpite. Nella stessa relazione emergono situazioni allarmanti. A partire dal 2010 la spesa sanitaria in Europa è diminuita per la prima volta da decenni. In Irlanda e Grecia i tagli alla spesa hanno superato il 6 per cento, invertendo un decennio di crescita con impatti negativi sulla salute pubblica. Nel *dossier* della Caritas italiana «Gioventù ferita», pubblicato nel gennaio 2015, si legge che in Grecia, per l'impossibilità di garantire un futuro ai propri ai figli, gli abbandoni dei bambini sono aumentati del 336 per cento negli ultimi cinque anni. Preoccupanti sono i dati della mortalità infantile. Questi sono i dati del vostro Governo. In Italia una donna su quattro rinuncia a prendersi cura di sé per dedicare i soldi alle spese per la famiglia. È questo il vostro amore per le donne. È quanto emerge dal volume «La salute delle donne: analisi e strategie di intervento», curato dall'Osservatorio nazionale sulla salute delle donne. Si tratta di una situazione non solo italiana: un quinto delle donne europee sviluppa un tumore prima dei settantacinque anni e quasi un terzo potrebbe essere individuato con la prevenzione e la riduzione dei fattori di rischio. Non voglio prolungarmi in queste celebrazioni, che non amo. Vorrei da questo Parlamento un'azione concreta nei confronti non delle quote rosa, non dei numeri, non delle donne messe lì tanto per fare numero, perché poi quando quando c'è un padre padrone, una madre padrona, un essere padrone è buon gioco ammettere le donne nelle posizioni di potere come delle controfigure. Vorrei ricordarvi che, al di là di tutti i vostri buoni propositi sulle quote rosa, in queste amministrative su quaranta candidati sindaci di tutti i partiti

delle maggiori città. Nel Movimento 5 Stelle, quando si lascia libertà ai cittadini, quando nessuno deve rimanere indietro e quando si hanno le mani libere per scegliere, non c'è bisogno di distinguere tra uomini e donne, perché saranno elette le persone che più rappresentano i cittadini, uomini o donne che siano.

tutte quelle donne coraggiose che cambiarono la storia, o meglio diedero inizio a un cammino di cambiamento in tema di giustizia e di diritti civili. In questi giorni, grazie anche a un famoso film, si parla della cosiddetta lotta delle suffragette, un termine che voglio ricordare essere spregiativo col significato: «ma dove vogliono andare queste?». Dico ciò perché sono parole ricorrenti tutt'oggi, di fronte ad ogni legittima ambizione delle donne. Dicevo, la lotta delle suffragette non fu solo una testimonianza culturale e intellettuale, ma una dura battaglia politica, che giunse anche a forti atti dimostrativi. Questo significa che la conquista dei diritti non fu facile nemmeno in un Paese come la Gran Bretagna, dove il pieno diritto di voto per le donne arrivò nel 1928, e in Italia solo circa vent'anni dopo. Ma il cammino per la parità dei diritti è stato tortuoso e difficile, e lo è tuttora, perché i cambiamenti culturali non seguono mai il passo dei cambiamenti legislativi. Non basta una legge, pur assolutamente fondamentale, per cambiare la mentalità e la cultura di un Paese. Non sono bastati settant'anni perché le donne raggiungessero davvero una piena parità dei diritti. C'è ancora molto maschilismo nella nostra cultura, nel nostro Paese; lo si respiro - ahimè - anche in quest'Aula, anche adesso, ogni giorno, anche se in un modo più subdolo e dunque, a parere mio, ancora più vigliacco. E al maschilismo purtroppo a volte si aggiunge anche - lo dobbiamo ammettere, noi donne - un'autoghettizzazione nostra, che spesso oscilla tra un femminismo ideologico e una sudditanza nei confronti della cultura dominante maschile. Noi donne dobbiamo liberarci dell'una e dell'altra posizione confidando più in noi stesse, non in quanto donne, ma in quanto persone, esseri umani. Il raggiungimento pieno della parità dei diritti è legato soprattutto al problema dell'educazione nelle famiglie e nelle scuole, e purtroppo su questo il nostro Paese mostra ancora molte lacune. Perché il punto vero - lasciatemi dire - è questo: i temi che riguardano i diritti civili e il raggiungimento della loro parità sono importanti non solo per chi non li vede riconosciuti in parte o appieno, non sono importanti solo per le donne o solo per gli omosessuali, ma sono importanti per tutti, anche per chi vive una posizione di privilegio. È importante capire questo, perché un Paese in cui vi è giustizia sociale, pari diritti e pari opportunità è un Paese capace di crescere, è un Paese capace di dare valore al merito, è un Paese capace di dare un futuro dignitoso a tutti. In conclusione, è un Paese migliore per tutti. Salutiamo gli studenti e i docenti dell'Istituto di istruzione secondaria «Luigi De' Medici» di Ottaviano, in provincia di Napoli, che stanno assistendo ai nostri lavori.

come hanno ricordato le mie colleghe - il 10 marzo del 1946 veniva concesso il diritto di voto alle donne. Fu un fatto storico importante, che ha rappresentato una tappa fondamentale per la costruzione dell'idea di cittadinanza definita dalla nostra Costituzione. Dopo gli anni bui del fascismo e della guerra, furono le vite e il sacrificio degli ultimi, degli operai, dei contadini, dei lavoratori, degli intellettuali, ad animare la resistenza come momento di riscatto e rinascita democratica. Un ruolo di primo piano lo ebbero le donne, protagoniste di una battaglia per la libertà in un momento drammatico della nostra storia. Raccontare alle ragazze e ai ragazzi di oggi che le donne, fino a settant'anni fa, non potevano votare, è un po' come parlare con loro della preistoria. 10 marzo di settant'anni fa vi fu la conquista dei diritti politici, che non fu, come spesso è raccontato velocemente nei libri di storia oggi, una concessione o un'estensione dei principi democratici, ma fu il risultato di una dura e lunga battaglia che fecero in prima persona le donne e non solo. La battaglia per la parità di accesso alla sfera pubblica, quella sfera pubblica che era stata costruita, nei secoli e nei millenni, proprio con l'esclusione delle donne, era legata strettamente alla battaglia di emancipazione dal ruolo di madre e moglie, da un ruolo secondario nella società. Non fu un caso che per la prima volta le donne parteciparono al voto, quel 10 marzo, per le elezioni amministrative, con un'affluenza oggi impensabile: l'89 per cento. Vennero elette oltre 2.000 candidate nei Consigli comunali, per lo più nelle liste della sinistra. Le donne dunque si fecero carico della vita pubblica, della vita sociale, della vita delle proprie città, dei propri paesi, dei propri concittadini; e smentirono così chi pensava che le donne italiane non fossero pronte a prendere parte alla vita democratica del Paese. Le 21 donne elette all'Assemblea costituente (su 156 deputati) furono determinanti per scrivere la nuova Costituzione e i suoi principi di uguaglianza e parità. Fu la socialista Merlin che - ricordo - fece inserire la parità di genere nell'articolo 3 e ancora tutti ricordiamo il ruolo di Teresa Mattei (tra l'altro, tra pochi giorni, è il terzo anniversario della sua morte), un ruolo fondamentale dell'articolo 3 della Costituzione; il suo «di fatto» ha reso l'articolo 3 un imperativo categorico per l'uguaglianza. La battaglia sul diritto di voto andò oltre e consentì di aprire la strada ad importanti ma faticose conquiste per la libertà e i diritti delle donne; anni durissimi di lotte, che coinvolsero tutti e tutte, i partiti, i sindacati, la società tutta. Furono importanti lotte per l'accesso al mondo del lavoro e il riconoscimento di diritti sociali e di libertà; anni lunghi, segnati anche da grandi sconfitte e da battaglie ancora da fare e per niente semplici. Oggi, con grandi responsabilità della mia generazione, si rischia di dare un po' tutto per scontato. Rischiamo di perdere la memoria, ma soprattutto di essere assuefatti ad un sistema che oggi, invece, registra numerosi passi indietro rispetto al tema della parità. Dunque spetta a noi, che stiamo ricoprendo questo importante ruolo istituzionale, raccogliere il testimone e riprendere il filo della parità ancora tutto da tessere. Non vorremmo incappare nella solita ritualità delle celebrazioni. Se ha un senso la nostra discussione oggi, è perché potremmo forse utilizzare questo nostro confronto per assumere degli impegni e, soprattutto, per impegnarci a rispettarli in maniera trasversale, anche se le logiche di partito e di appartenenza indicheranno di fare altro e prendere altre strade. Questo, d'altronde, fu lo spirito delle donne che lottarono per il riconoscimento del diritto di voto e questa la scelta politica delle donne dell'Assemblea costituente. Potremmo fare una lista dei nostri futuri prossimi impegni: parità di presenza nelle liste elettorali, parità sempre quando si devono indicare quote (non più 60 e 40 per cento, ma coraggiosamente 50 parità di accesso al lavoro, parità salariale, misure a tutela del *welfare* familiare, libertà di scelta (ad esempio, no ai medici obiettori nel servizio pubblico), tutela della salute delle donne, in particolare nei luoghi di lavoro. Ad esempio, il senatore Barozzino racconta sempre della condizione di lavoro delle donne in tuta bianca nelle fabbriche di Melfi e su questo potremmo forse cominciare a dare indicazioni concrete. lotta contro la violenza di genere e l'assunzione di tutte le precarie della scuola pubblica. Certo, si tratta di una lista parziale da integrare, ma ciò che è importante è il patto che facciamo tra noi trasversalmente: questa sarebbe la novità.

perché è bene che questa battaglia, che ha aperto la strada a ben altre conquiste, possa essere patrimonio di tutti. Vorremmo soprattutto cominciare il lavoro per la parità a partire dalle scuole, perché sappiamo che la lotta contro le discriminazioni e per la parità deve partire da lì. Avevo notato tra le file del Governo la presenza della sottosegretaria D'Onghia e pensavo potesse essere un argomento da inserire nei vari POF della scuola. Potrebbe essere interessante, perché si tratta di un lavoro che deve coinvolgere tutti: bambine e bambini, ragazzi e ragazze,

scriveva: «Tra i giornalisti ci fu un moto che si potrebbe chiamare di sfiducia preventiva. Molti politici vennero presi dall'impellente desiderio di bersi un caffè, altri andarono a fumare nei corridoi, riaffacciandosi di tanto in tanto per scambiarsi sottovoce frasi non troppo nuove sulle pentole che l'oratrice avrebbe fatto bollire e sulle calzette che non aveva potuto rammendare». Non vorrei che oggi ci trovassimo in quella stessa situazione.

delle istituzioni a celebrare la Giornata internazionale della donna. Il Senato arriva a tale appuntamento in questo modo, dal mio punto di vista sbagliato, perché non coordinato e concertato soprattutto tra quelle parlamentari, cioè tutte noi, che più si fanno carico di sostenere l'azione in Parlamento, rifacendosi alla storia di quelle donne che votarono per la prima volta e alla storia di alcune particolari donne che, elette in Assemblea costituente, diedero uno straordinario contributo. Vorrei ricordare una frase di Teresa Mattei, che è stata appena citata. È molto cara a tutte noi donne, anche se di orientamenti politici diversi. Diceva: «Noi non vogliamo che le nostre donne si mascolinizzino, non vogliamo che le donne italiane aspirino ad un'assurda identità con l'uomo; vogliamo semplicemente che esse abbiano la possibilità di espandere tutte le loro forze, tutte le loro energie e tutta la loro volontà tutta la loro volontà di bene nella ricostruzione democratica del nostro Paese». Lo dichiarò nella seduta del 18 marzo del 1947. Era una di quelle 21 donne che segnarono con la loro cifra la Costituzione che abbiamo. Senza quelle donne non avremo nemmeno questa Costituzione, a partire dall'articolo 3, ampio e solido, scritto e voluto soprattutto da loro. Il percorso delle donne verso una piena cittadinanza cominciò. Ma in Italia è stato reso più tortuoso che altrove, non solo da una disomogeneità molto forte delle culture locali e regionali, ma anche dalla pesante influenza di una cultura che ha troppo a lungo favorito l'identificazione delle donne con la famiglia e la difesa dei lavori comunitari minacciati dai processi di modernizzazione. Così si diceva all'epoca. Infatti, sebbene il testo costituzionale rappresentasse nel suo insieme un progresso per le donne italiane, i limiti in esso contenuti sarebbero stati destinati a pesare fino ad oggi. L'articolo 37, infatti, nonostante attribuisse alle donne stessi diritti e uguale retribuzione dell'uomo a parità di lavoro, prevedeva: «Le condizioni di lavoro devono consentire alla donna l'adempimento della sua essenziale funzione familiare». Noi oggi siamo arrivati a completare questo pensiero, poiché tutto questo sta in capo agli uomini e alle donne che costituiscono una famiglia. È evidente la scollatura tra i desideri, i bisogni e le attese delle donne italiane del dopoguerra e la realtà, che vivevano e viviamo ancora oggi, poiché il voto non comportò la pienezza dei diritti politici e, soprattutto, non corrispose per molto tempo alla pienezza dei diritti civili. Il salario femminile per lo stesso tipo di lavoro, ad esempio, rimase sempre inferiore e nel 1954 la firma di un accordo sindacale che stabiliva solo cento la differenza salariale tra i lavoratori e le lavoratrici venne accolta come una vittoria. Come vedete, a distanza di tanti anni, oggi siamo ancora qui a discuterne, nonostante i numeri della formazione scolastica e universitaria che sono stati negli anni ribaltati totalmente dalle donne, a loro Anche sul piano occupazionale la situazione italiana era difficile (e lo è ancora oggi), sebbene non drammatica come nel primo dopoguerra. Le donne dovevano infatti difendere i loro posti di lavoro, anche contro il sindacato che tutelava fortemente i salari maschili e soprattutto le posizioni lavorative degli uomini. Questo accadde quando gli uomini rientrarono dal fronte. È finita la guerra; è scoppiata la pace; è cominciata la ricostruzione, ma, ancora una volta, le donne pagano il prezzo più alto. Oggi, invece, li devono difendere dalla flessibilità e dalla precarietà, che su loro pesa ancor di più a causa della mancata flessibilità di quello Stato e dei suoi servizi che continuano a impedire che nel nostro Paese si raggiunga una giusta ed equilibrata partecipazione femminile al mercato del lavoro lavoro e, come avviene negli altri Paesi, un incremento demografico degno di un Paese che non guarda solo al suo passato, ma anche al suo futuro. Il lento riconoscimento di fondamentali diritti, ottenuto grazie all'attivismo delle associazioni femminili che hanno permesso, con tenacia, un adeguamento legislativo che, pur tra resistenze e ritardi, avrebbe consentito di raggiungere almeno una parità giuridica formale, transitato da alcune importanti leggi, sostenute con forza dalle parlamentari donna, è un percorso ancora a metà. La cittadinanza femminile é rimasta e resta tuttora una cittadinanza debole, fatta di avanzamenti parziali e di attese tradite. Alla pienezza dei diritti politici delle donne non corrisponderà per molto tempo la pienezza dei diritti civili, acquisiti molto lentamente. Basti pensare che, da quel 1945, un po' alla volta, la donna si è conquistata un ruolo chiave, sia sul campo di battaglia che nelle fabbriche, sostituendo di fatto l'uomo, impegnato al fronte. Questo è ciò che avvenne durante la guerra. La legge di tutela delle lavoratrici madri è però del 1950 - ancora oggi è considerata una delle più avanzate d'Europa -, quella che consentiva per la prima volta l'ingresso delle donne nell'amministrazione della giustizia è del 1956, e quella che consentiva la costituzione della polizia femminile Il divieto di licenziamento per matrimonio è del 1963, 1'abrogazione dell'articolo sul diverso trattamento - ascoltatemi bene! - tra l'adulterio maschile e l'adulterio femminile è del 1968 la legge sul divorzio è del 1970. Anche all'interno della famiglia e nella società, con la riforma del diritto di famiglia del 1975, la condizione della donna è radicalmente mutata: è stata abolita la figura del capofamiglia e la donna e l'uomo hanno pari diritti e pari doveri, sia sulle decisioni che riguardano direttamente la coppia, sia sui figli. È del 1991 la legge n. 125 sulle azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro, alla faticosa approvazione, nel 2012, della legge Golfo-Mosca, sulle quote rosa nelle società a partecipazione pubblica e nelle società quotate. Ricordo che dobbiamo attendere il 1994

Solo nel 2009 viene introdotta la norma che considera reato l'odiosa pratica degli atti persecutori contro le donne e non solo, che va sotto il nome di *stalking*. Nel 2013 abbiamo dovuto inasprire le pene e le misure cautelari contro il femminicidio, proteggendo chi denuncia, per aiutare a far emergere, a far uscire spesso dalle mura domestiche i casi di violenza, che non vogliamo più accettare. attorno al ruolo femminile, tra elettorato passivo ed elettorato attivo, è ancora in corso, come hanno ricordato molte colleghe prima di me. Le leggi elettorali amministrative costituiscono un'azione positiva e forse - chi lo sa? - persino l'Italicum può essere considerato un piccolo passo in avanti, per riequilibrare una rappresentanza messa a dura prova dall'imbarbarimento della politica. Auguriamoci che quella legge elettorale non prosegua sulla strada dell'imbarbarimento della politica. In molti Paesi il voto alle donne non coincide con il riconoscimento di diritti civili e sociali e talvolta convive, quotidianamente, con la violazione dei diritti umani. Sono note a tutti le donne afghane o irachene che, velate, si recano alle urne, per rappresentare con forza il loro diritto. È evidente, dunque, che la storia del voto alle donne è strettamente legata, fin dalle origini, alla storia della democrazia e delle sue ridefinizioni, e dunque non si è ancora conclusa.

Ci sono studi di Banca d'Italia secondo i quali se l'occupazione femminile fosse al 60 per cento, come fissato dagli obiettivi di Lisbona, il nostro PIL crescerebbe del 7 per cento. Ma dall'altra parte del mondo ci sono ancora bambine costrette a sposare sconosciuti molto più vecchi di loro, a vendere il proprio corpo o a lavorare a piedi nudi per due soldi. Molte di quelle donne arrivano da noi, confuse tra i viaggi disperati di migliaia di esseri umani, destinate ad un futuro non migliore di quello da cui scappano, nel silenzio delle nostre città La condizione di queste donne, vittime della radicalizzazione dell'Islam, spesso anche nel nostro Paese, deve farci riflettere. C'è poi il divario, sempre più stridente, con ciò che accade ogni giorno sotto i nostri occhi, nei nostri Paesi e nelle nostre città: lo scorso anno, le donne uccise in Italia sono state 128. Soltanto nei primi 50 giorni di quest'anno si contano già 13 vittime. Sono quelle che non ce l'hanno fatta, ma infinitamente di più sono quelle che subiscono violenze fra le mura domestiche, senza denunciare, nell'assoluto silenzio. Ebbene, questa celebrazione sia soprattutto di quelle donne, perché non vi sono conquiste politiche, sociali ed economiche di cui andare fieri, fino a quando ci saranno discriminazioni e violenze su di noi.

Signor Presidente, le ruberò pochi secondi per ristabilire un minimo di equilibrio di genere, anche perché sono intervenute solo delle senatrici,

se, peggio ancora, qualcuno se ne è dimenticato (perché in quel caso sarebbe particolarmente grave), oppure se qualcuno consideri già chiuso questo ramo del Parlamento. Sono Sono convinto che se il Senato deve diventare ciò che è stato prefigurato dalla nostra riforma, tanto vale chiuderlo; tuttavia, finché c'è io apprezzerei che quella deriva, che nella discussione sulle riforme

passivo ai consiglieri regionali e lo abbiamo esteso anche ai sindaci al livello dei consiglieri regionali. Visto il numero di consiglieri regionali attualmente presenti nel nostro Paese, oggi stiamo festeggiando un diritto che giustamente è stato attribuito alla la donna è meno rappresentata che in altre sedi.

Con quello che sta accadendo, limitare il voto per il Senato a determinate categorie, non vorrei che in futuro qualcuno limitasse il voto anche ad altre categorie.

preavvertire il Senato per avere una partecipazione più attenta; dopo di che, così si è deciso, e da questo punto di vista anche alcuni Gruppi hanno sottolineato che una programmazione dei lavori avrebbe

dagli inizi degli anni Sessanta è attivo lo stabilimento produttivo sartoriale del marchio Brioni, che oggi conta oltre 1.200 dipendenti. La produzione di abbigliamento di lusso per uomo e di capi su misura è conosciuta in tutto il mondo per la pregiatissima qualità che porta il marchio stesso ad essere un *leader* mondiale. La lungimirante politica aziendale ha portato l'azienda ad inaugurare nel 1985 una scuola di sartoria proprio a Penne con l'obiettivo di trasmettere il metodo sartoriale Brioni alle nuove generazioni di sarti. Attualmente in Abruzzo sono presenti stabilimenti produttivi tutti concentrati nell'area Vestina (quindi Penne, Montebello di Bertona e Civitella Casanova) e - come già detto - ci sono circa 1.200 lavoratori. Tra il 2011 e il 2012 la Brioni viene acquisita dal gruppo francese Kering che ne modifica le caratteristiche produttive che portano a scelte industriali diverse dalla sua tradizione artigianale. A causa di crisi dovute a commesse mancate, probabilmente, ed anche ad un'errata politica industriale che ha cercato di mutare il caratteristico stile Brioni, l'11 novembre 2015 è stata firmata l'apertura della mobilità volontaria, che resterà aperta fino al 31 dicembre 2016, per 50 lavoratori. La crisi di commesse, però, ha portato l'azienda ad una sovrapproduzione di capi, tant'è che in questi giorni ha annunciato un probabile esubero di 400 posti di lavoro. La Brioni, oltre ad essere la più importante realtà produttiva industriale dell'area vestina della provincia di Pescara, detiene un patrimonio sartoriale unico e prezioso. La crisi aziendale, preannunciata e ipotizzabile con largo anticipo, porterebbe inevitabilmente ad una crisi economica e sociale molto grave nella provincia di Pescara. La crisi aziendale è talmente sentita a livello locale che l'assemblea pubblica, scaturita dall'annuncio della riorganizzazione aziendale con esubero di 400 posti di lavoro, ha riempito gli spalti dello stadio comunale di Penne. Quindi, chiedo oggi qui con forza ai Ministri del lavoro e dello sviluppo economico di distogliere l'attenzione da lobbysmi vari e da richieste di multinazionali e di iniziare a pensare davvero agli imprenditori, quelli veri, e ai lavoratori, assumendo immediatamente iniziative per affrontare la crisi industriale della Brioni, anche promuovendo tavoli di confronto con la proprietà dell'azienda, le parti sociali e le istituzioni regionali abruzzesi, con il fine di tutelare i livelli occupazionali e la tradizione artigianale sartoriale. *(Applausi

di attenzione e iperattività o ADHD, indirizzata al ministro della salute Lorenzin, presentata da quasi due anni, il 13 marzo 2014, link apre una nuova finestra") per un riscontro che spero ora sia maggiormente tempestivo. L'ADHD è un disturbo evolutivo dell'autocontrollo che si manifesta con difficoltà di attenzione, concentrazione e controllo degli impulsi. L'ADHD World Federation classifica l'iperattività infantile come «una malattia altamente ereditaria, della quale soffrirebbe il 5 per cento dei minori nel mondo, bambini ed adolescenti che sarebbero potenziali destinatari di terapie a base di anfetamine». Molto spesso in Italia però, in ambito soprattutto scolastico, si confonde la normale distrazione e vivacità dei minori con il vero e proprio disturbo ADHD testé menzionato, senza tenere conto che alcuni comportamenti dei minori sono direttamente ascrivibili alla noia derivante da attività scolastiche non adeguate ai tempi di apprendimento dei ragazzi oppure alle difficoltà emotive correlabili a situazioni di particolari disagi per crisi familiari, mal gestiti o addirittura amplificati a seguito di inopportuni allontanamenti del minore dalla famiglia d'origine, come sta emergendo nelle audizioni dell'indagine conoscitiva sui minori fuori famiglia che ho promosso in Commissione infanzia e adolescenza. Le cause dell'ADHD non sono ancora del tutto ben definite e uno studio condotto dall'università di ha rilevato un legame diretto tra ADHD e maltrattamenti fisici subiti dai bambini. Si riscontra pertanto una notevole leggerezza del personale medico nel diagnosticarlo, con conseguente diffuso intervento farmacologico. A tal proposito, l'utilizzo di farmaci anfetaminici come il Ritalin ha evidenziato un peggioramento delle funzioni mentali, l'impoverimento della creatività e la perdita di emotività da parte di bambini ed adolescenti. Per tutto questo tempo - sono anni - non ho avuto nonostante il numero di visite per ADHD sia notevolmente aumentato su tutto il territorio nazionale e non soltanto nelle province di Teramo e Pescara. Chiedo, pertanto, al ministro Lorenzin di fornire il numero esatto di tutti i bambini sottoposti a diagnosi e trattamento farmacologico per sindrome di ADHD, con particolare riguardo alla Regione Abruzzo, e di chiarire le eventuali iniziative che intende porre in essere per individuare un serio percorso diagnostico e per rispondere agli studi e alle istanze di numerosi istituti, specialisti specialisti e associazioni come l'INPEF, che utilizzano un approccio metodologico e didattico con ottimi risultati.